il Consiglio presidenziale presieduto dal *premier* al-Sarraj si è insediato il 30 marzo scorso a Tripoli. Questo evento, lungamente atteso non solo dall'Italia e dalla comunità internazionale, ma soprattutto dalla popolazione libica, ha rappresentato senza dubbio un avvenimento importante politicamente, ma soprattutto di grande valore simbolico. il 12 aprile scorso, lei si è recato, primo tra i rappresentanti di un Governo straniero, nella capitale per incontrare il *premier* al-Sarraj e il Consiglio presidenziale. Sappiamo bene che ci troviamo all'inizio di un percorso lungo e difficile, che ha anche in sé un ambito di fragilità molto evidente, il controllo della capitale continua a rappresentare una sfida assai rilevante per le nuove autorità che sono chiamate ad affrontare la situazione di quel Paese. La situazione nell'est della Libia resta, tuttavia, molto preoccupante. All'interno della Camera dei rappresentanti di Tobruk vi è una solida maggioranza a favore dell'Esecutivo, ma alcuni personaggi continuano a impedire un regolare voto di fiducia attraverso intimidazioni e minacce nei confronti di questi parlamentari.

dalle notizie di stampa - per le installazioni petrolifere e il rischio che con la buona stagione si accentui il fenomeno di partenza di profughi dalle coste libiche inducono preoccupazione. Alla luce di questa situazione,

Signor Presidente, nel pochissimo tempo che ci è consentito porrò tre domande velocissime. La prima. Vorremmo sapere qual è lo stato di avanzamento di EUNAVFOR Med, che molti dicono debba passare alla terza fase; siamo fermi alla seconda fase e mezzo e vorremmo sapere se siamo nelle possibilità, con l'accordo di tutti i Paesi europei o, per lo meno, di coloro che vi partecipano, di passare alla fase tre, che prevede anche la possibilità di bloccare i barconi prima della partenza. Il secondo quesito riguarda il generale Haftar, che è un grande ostacolo al processo di stabilizzazione della Libia. Haftar, il Governo e il Parlamento di Tobruk vantano il fatto di aver liberato l'80 per cento di Daesh e tutto sommato questa è stata un'operazione militare che va nella direzione auspicata dalla comunità internazionale. Tuttavia, questo vuol dire che l'esercito del generale Haftar è nelle condizioni di combattere efficacemente Daesh anche in altre città nella fattispecie, vorrebbe andare a Sirte, che, però, è nella parte riservata, teoricamente, al Governo di Tripoli. Siccome mi sembra che la presenza ingombrante del generale Haftar, soprattutto per l'ottenimento della fiducia da parte del Governo di Tripoli, sia tale da rendere impossibile, alla fine,

a sua informazione, sa se qualche Paese europeo, prima che venga definita la famosa missione internazionale a guida italiana, abbia per caso intenzione di

Grazie, signor Presidente. Buon pomeriggio, signor Ministro. prevedeva l'approvazione del Governo con voto di fiducia da parte dell'House of representatives, ma, ad oggi, questo voto di fiducia ancora non vi è stato. UNSMIL descrive Tripoli come una realtà frammentata, con presenza di forze filogovernative o oppositrici. Ci sono circa 41 gruppi armati, dei quali l'80 per cento supporta il Government of national accord (GNA), ma solo nell'area pro-GNA ci sono circa 12 forze o gruppi armati e anche a Bengasi la situazione sembra molto simile a quella di di Tripoli. Nelle stesse ore, però, il Governo italiano presenta in Europa il *migration compact*, cioè una serie di intenti per gestire e contenere i flussi migratori, con un capitolo speciale proprio dedicato alla Libia. Il *migration compact* parte libica non sembra, però, aderire allo scenario descritto e proposto da UNSMIL, risultando quindi di difficile attuazione, proprio perché non coerente con la situazione a terra. Il fenomeno migratorio assume, dunque, un ruolo centrale, che molti indicano come merce di scambio tra interessi diversi. Nel 2015, 154.000 migranti arrivano nell'Unione europea attraverso la Libia e, nel 2016, su 5.270 arrivi il 97 per cento proviene proprio dalla Libia. Per questi motivi, le chiedo se e su quali temi il Governo abbia interagito con l'ONU-UNSMIL per la redazione del *migration compact*, parte libica, per la corretta valutazione della posizione italiana circa un probabile intervento militare di terra in Libia e delle possibili conseguenze, anche alla luce di quanto indicato da alcuni analisti, secondo i quali ISIS attacca maggiormente se attaccato o comunque costretto ad arretrare in quello che considera il proprio territorio. Infine, vorrei sapere se ritiene che la richiesta di assistenza rivolta all'Italia dovrebbe essere valutata solo dopo aver verificato il sostegno al-Sarraj, che sarebbe allora un Governo di rappresentanza nazionale di autodeterminazione del popolo libico e, a quel punto, valutare anche la riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli. [DI con riferimento all'evoluzione della crisi in Libia, credo sia un'opinione sempre più condivisa l'auspicio di una soluzione unitaria con il riconoscimento da parte di tutti del Governo di unità nazionale e quindi il suo consolidamento, condizione imprescindibile per stabilizzare quell'area. Appare però ormai evidente come uno degli ostacoli a questa soluzione sia rappresentato anche dalla figura dell'ex generale Khalifa Haftar, capo delle Forze armate di Tobruk. Il generale viene sostenuto economicamente, diplomaticamente e militarmente dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Egitto, i quali, nonostante l'embargo, forniscono alle truppe strumenti, armi e sostegno finanziario. Vale la pena ricordare che nei giorni scorsi sono approdati nel porto di Tobruk un migliaio di veicoli da combattimento insieme ad armi e munizioni, che lasciano presagire le potenzialità e le mire strategiche in Cirenaica, soprattutto sul versante del controllo dei pozzi petroliferi. Tutti noi siamo consapevoli dei risvolti strategici geopolitici di tale eventualità, avanzata contemporaneamente non soltanto in termini di stabilità territoriale, ma anche nello scacchiere internazionale. Ovviamente questa fornitura, illegittima se si considera l'embargo, appare collegabile alla coalizione panaraba che sostiene Haftar. In questo scenario, considerando le posizioni dubbie che sta assumendo il Governo francese nei confronti di Haftar, che sostanzialmente non sembra essere in linea con quelle europee, sarebbe auspicabile conoscere la posizione ufficiale del Governo di Parigi rispetto alla crisi libica, considerando la posizione contraddittoria che lo sta condizionando, quali siano i rapporti effettivi della Francia con l'ex generale Haftar e se vi siano effettivamente dei coinvolgimenti di carattere militare.

spesso smentite, di allusioni e anche di interviste rilasciate da esponenti del Governo che alludono all'invio di militari italiani in Libia. In genere non si parla di guerra, anche se mi chiedo cos'altro sia un intervento armato in un Paese che è in guerra, ma quello che vorrei chiederle, signor Ministro, è: contro chi e a favore di chi. Contro Daesh? Ma anche contro il generale Haftar? Abbiamo visto la bandiera italiana bruciata in piazza ieri. Sappiamo che il generale Haftar ha l'appoggio dell'Egitto, che vuole combattere l'ISIS, il Daesh, ma anche i Fratelli musulmani e che è ostile al Governo che si è insediato a Tripoli. E poi le chiedo, signor Ministro: le milizie islamiche che stanno appoggiando detto Governo le consideriamo degli alleati? Ci fidiamo di loro o no? Inoltre, signor Ministro, si dice spesso che questo intervento sarebbe meno rischioso e grave, perché si tratta non di fare una guerra offensiva contro Daesh, ma di difendere sedi a Tripoli o addirittura pozzi nel deserto.

dibattito su una cosa che non prevedeva l'invio di soldati sul campo, cioè i bombardamenti in Siria. Quando il Governo si deciderà a chiedere una sessione del Parlamento che discuta a fondo di questa questione? Signor Presidente, signor Ministro, tutti conosciamo l'importanza che la Libia ha, per un fatto strategico, nei confronti dell'Italia. Però, proprio per questo, nel momento in cui il Consiglio presidenziale libico e il presidente al-Sarraj si sono insediati, sono ancora senza un voto di fiducia da parte del Parlamento riconosciuto dalla comunità internazionale, che è quello di Tobruk. Accanto a questa situazione vi sono degli episodi, alcuni dei quali citati.

del Consiglio presidenziale libico, di bloccare l'offensiva di Haftar per quanto riguarda Sirte, che lo stesso Haftar ha esaltato ricordando una battaglia del 1915 contro l'Italia. Di fronte a questa situazione, c'è una dichiarazione dell'ambasciatore della Libia Santa Sede, che pare abbia chiesto all'Italia protezione per le ambasciate e per le sedi ONU e addirittura un coinvolgimento italiano in difesa dei confini libici, sia in terra che in mare e si parla anche di una dichiarazione del ministro Pinotti di un intervento della NATO. Su questo vorremmo avere notizie da parte del Governo. [MAURO

regionale, così anche in Libia ci sono Paesi influenti che in questi giorni, da molti mesi, da alcuni anni, determinano le sorti di quello che accade sul terreno. Uno è già stato citato ampiamente dai colleghi, l'Egitto, mentre l'altro è la Turchia; il rapporto di*leadership* che il premier Erdoğan ha intrapreso all'interno della Fratellanza musulmana ne fa stabilmente un punto di riferimento non solo per chi governa a Tripoli, ma anche per le ambigue e a volte apparentemente contraddittorie prese di posizione degli alleati occidentali. già è emerso dagli interventi dei colleghi, ci si chiede: chi sta con chi? Chi fa gli interessi di chi? Da questo punto di vista, quali sono le scelte strategiche dell'Italia, anche rispetto al ruolo di Egitto e Turchia in Libia?

con due grandi fori, se uno è stato tappato, quello della rotta balcanica, meno si sa di quello che potrà accadere per la rotta libica. Le chiedo allora: nella messa a punto dell'accordo tra Unione europea e Turchia è stato previsto qualcosa che, indipendentemente dalle proposte successive e forse tardive del *migration compact*, sia elemento di sicurezza, cerniera e chiusura anche del fronte libico?

nazionale, dell'arrivo in Libia del *premier* al-Sarraj, designato dal Governo di accordo nazionale. Ci hanno anche descritto le modalità del suo arrivo, non senza screzi e addirittura tra qualche sparo. sparo. Sembra che il *premier* al-Sarraj si trovi ancora presso una base navale, sempre nei pressi del porto di Tripoli e questo ci lascia intuire che il nuovo Governo non è proprio in grado di assumere, almeno per ora,

al-Sarraj adesso chiede alla comunità internazionale, a noi e all'Europa tutta, un intervento militare, innanzitutto con lo scopo di sradicare l'ISIS dalla Libia, ma anche, e non ultimo, con quello di proteggere le infrastrutture dell'industria petrolifera da potenziali attacchi di miliziani e di jihadisti che fanno riferimento al califfato. Questa operazione sembra che sia benedetta o comunque veda di buon grado,

Secondo lei, signor Ministro, quali prospettive ha il Governo di al-Sarraj di riuscire a consolidarsi in questo contesto, visto che è ancora vincolato in una base navale? Cosa intende fare l'Italia per sostenerlo, soprattutto dal punto di vista militare?

che un chiarimento definitivo sul numero verrà dato, se e quando sarà necessario, in Parlamento e senza che il Presidente del Consiglio debba svolgere ogni settimana una sorta di funzione di addetto stampa del Governo per «frenare», come si legge sui giornali. Il punto è che nelle cronache di politica internazionale che, a differenza del nostro Paese, da parte di altri Paesi europei, in particolare della Francia, si dia per irrimediabilmente perduta, compromessa e non recuperabile l'unità statuale libica. Senza ricorrere nazionalisticamente al ricordo di come questa unità dello Stato libico sia stata a suo tempo frutto e opera italiana (non dell'Italia fascista ma dell'Italietta liberale), a me sembra che sia necessario che l'Italia, al di là dei numeri del contingente militare (se, come e quando sarà), chiarisca se opera per la ricostruzione dell'unità statuale in Libia o soltanto in funzione di protezione e garanzia di questo o quel Governo.

molti onorevoli senatori hanno espresso preoccupazione e dubbi sulla possibilità che il processo in corso in Libia possa essere lineare

Sappiamo tutti molto bene quale sia la difficoltà e la fragilità del processo in corso, e purtroppo sotto sotto il titolo «fragilità» potremmo racchiudere non solo la Libia, ma molte delle crisi internazionali nel Mediterraneo e in altre aree con le quali abbiamo a che fare. Il punto è se la direttrice di marcia in cui ci muoviamo è corretta e se ha margine di attuabilità, e credo che questo si possa dire, con tutta la premessa della fragilità, di come ci stiamo muovendo in Libia. Abbiamo fatto un'operazione diplomatica nel mese di dicembre, con una conferenza che in un certo senso è stata il trampolino di marcia di un accordo che si è concluso due giorni dopo in Marocco e di una risoluzione dell'ONU che è stata adottata quattro giorni dopo a New York. Su quella base è nato un Governo di intesa nazionale. Sembrava molto difficile, nei primi mesi di quest'anno, che riuscisse non dico a stabilizzare la Libia, ma addirittura a non essere un Governo in esilio: era un Governo a Tunisi, si è stabilito il 30 marzo a Tripoli. È in una situazione stabile a Tripoli? Certamente no: è in una situazione fragile. È vero che il presidente al-Sarraj è tuttora nella base navale del porto, ma è altrettanto vero che sette o otto ministri hanno preso possesso dei loro Ministeri a Tripoli, e che la situazione a Tripoli e nell'area fra Tripoli, Misurata la Tripolitania in genere, è relativamente sotto il controllo della maggioranza delle milizie e delle forze ufficiali fedeli a questo Governo. Avendo verificato che Avendo verificato che sono stati fatti dei passi in avanti, ma che questi passi restano tuttora fragili, in che direzione va il lavoro che dobbiamo fare? Con la premessa che ha ricordato il senatore Compagna e cioè che noi siamo sempre stati e siamo per il mantenimento dell'unità della Libia. Qui non si tratta di discettare sulla correttezza o meno degli accordi Sykes-Picot o sulla natura storica o meno della Libia. Qui stiamo parlando di di politica e di assetti strategici: la frantumazione di un Paese come la Libia sarebbe una minaccia geopolitica per l'intero Mediterraneo e per l'Europa; il mantenimento della sua unità è nel nostro interesse.

in che misura lo si può fare. Certamente, sarà utile se la maggioranza della Camera dei rappresentanti di Tobruk, che finora si è espressa firmando dei documenti e non con una seduta, potrà dargli una fiducia

le armi non embargate (vale a dire quelle per combattere il terrorismo) e il commercio del petrolio devono far capo al Governo legittimo d'intesa nazionale. Stanotte il Comitato sanzioni delle Nazioni Unite ha listato la nave battente bandiera indiana, ma di proprietà - credo - emiratina, che aveva caricato un numero molto consistente di barili di petrolio dalla dalla Libia e si stava dirigendo verso Malta. In secondo luogo, occorre evitare spinte centrifughe. Tutti devono essere coinvolti nel processo.

Nei confronti di queste tre persone l'Unione europea ha deciso sanzioni. Una di queste tre persone, cioè al-Gwell, è anche sanzionata dagli Stati Uniti. Il resto, cioè le persone che non sono oggetto di sanzioni, possono avere posizioni più o meno condivisibili, ma se noi lavoriamo in un'ottica di di riunificazione della Libia, dobbiamo fare ogni sforzo per coinvolgerle nel processo, altrimenti parliamo di riunificazione della Libia ma in realtà alimentiamo tendenze alla sua divisione. Oggi, infatti, la nostra preoccupazione principale è la nascita di spinte centrifughe che possano mettere in discussione l'unità del Paese. In terzo luogo, dobbiamo lavorare per aiutare il Governo nella stabilizzazione, rapporti bilaterali di vario tipo. Non siamo solo stati i primi ad andare in visita al Governo a Tripoli, stiamo ricevendo continuamente delegazioni di Ministri di questo Governo e stiamo avviando collaborazioni; sul piano umanitario, nei prossimi

Verrà anche il giorno in cui, se il Governo libico lo riterrà, se si considererà sufficientemente forte per fare delle richieste sul terreno del *training* delle proprie forze di sicurezza, ci potranno anche essere compiti su tale terreno, ma abbiamo ripetuto (e lo faccio ancora una volta, facendo anche io l'addetto stampa di me stesso) che noi daremo questo contributo sulla base delle richieste del Governo libico e di una validazione delle Nazioni Unite. Per ora queste richieste non ci sono state, neanche sul terreno, di cui pure molto si è parlato sui giornali, della protezione dei pozzi petroliferi. Il Governo libico ha diramato un comunicato stampa richiamando la comunità internazionale al rispetto della risoluzione n. 2278 delle Nazioni Unite, non ha mandato una lettera agli italiani, ai francesi, agli americani o agli inglesi chiedendo l'invio di truppe, come è parso essere presentato quel comunicato stampa.

una superpotenza, ma siamo certamente un Paese determinante in questo campo: in tutti i consessi, dall'Unione europea al G7, quando si parla di Libia è l'Italia che illustra e propone una visione e una posizione.La posizione è quella di cui ho detto: stabilizzazione di un Paese unito e graduale risposta a eventuali richieste, all'inizio umanitarie, poi verranno quelle economiche quando si sentiranno sufficientemente robusti, verranno anche quelle sul terreno della sicurezza. In questa prospettiva non possiamo fare processi alle intenzioni. Dal punto di vista delle posizioni politico-diplomatiche, se interrogate la diplomazia egiziana o quella francese vi diranno che sono assolutamente su questa lunghezza d'onda e sostengono il Governo

Italia e Stati Uniti lavoreranno nelle prossime settimane per rilanciare questo concerto diplomatico a sostegno del percorso del Governo al-Sarraj, perché forse c'è bisogno di un richiamo, di un *refill*, di un rilancio di un *refill*, di un rilancio di questo concerto diplomatico a sostegno del Governo. Infine, due elementi fondamentali in questo percorso, che molti dei senatori interroganti hanno sollevato, riguardano, da un lato, il tema migrazioni e, dall'altro, il tema contrasto al terrorismo. Sul tema migrazioni è chiaro che siamo tutti a favore - ne abbiamo discusso in un recente Consiglio esteri-difesa dell'Unione europea - del passaggio alla fase successiva della missione EUNAVFOR Med, di cui ha parlato il senatore Romani. È altrettanto chiaro che, com'è scritto nella nella decisione del Consiglio europeo che l'ha istituita, per il passaggio alla fase tre serve una richiesta delle autorità libiche. Per ora questa richiesta non è arrivata, perché la fase tre, come sapete, comporta innanzitutto l'ingresso in acque territoriali libiche. In qualche modo la stiamo sollecitando, ma dobbiamo stare molto attenti a non dare, anzitutto al popolo libico, l'impressione che le autorità libiche siano delle autorità manovrate dall'esterno. Quando diciamo che il primo obiettivo è il consolidamento, vuol dire che bisogna affermare una rappresentanza libica di questo percorso. Se le autorità libiche apparissero manovrate dall'esterno il loro consolidamento sarebbe molto problematico. Quindi, certamente ci vuole la fase tre, ma a mio parere occorreranno alcune settimane prima che le autorità libiche si possano ritenere sufficientemente consolidate da poter fare domande di questo o di altro genere alla comunità internazionale. Intanto noi, in sede bilaterale, ne stiamo discutendo. Il Ministro degli interni è venuto al Viminale qualche giorno fa. Il *migration compact* non è indirizzato alla Libia e non possiamo autorizzare alcun paragone tra Libia e Turchia. La Turchia è un Paese sovrano, addirittura definito Paese sicuro per il rientro dei migranti ed è stato fatto un certo tipo di accordo. Non possiamo immaginare lo stesso accordo con la Libia. Possiamo però bilateralmente cooperare e, sul piano multilaterale, EUNAVFOR Med e il riposizionamento di Active endeavour, cioè della missione NATO, possono dare una mano a gestire il Mediterraneo dal punto di vista dei flussi. Infine, per quanto riguarda il tema del terrorismo,

Molti tra i libici definiscono i terroristi di Daesh come stranieri. Per loro sono gli stranieri. C'è una singolare competizione, oggi, tra diverse componenti del frastagliato panorama libico, per chi combatte contro Daesh e per chi, prima dell'altro, va a intervenire su Sirte. Se scavalcassimo queste dinamiche con un intervento esterno, a mio parere faremmo un grave errore. Peraltro è escluso che possano farlo singoli Paesi europei, dato che, come sappiamo benissimo, per compiere interventi antiterrorismo di una certa consistenza senza la partecipazione attiva degli Stati Uniti e il controllo che gli Stati Uniti hanno, da mille punti di vista, in quell'area, un singolo Paese europeo non va lontano e sappiamo che gli Stati Uniti hanno finora condotto soltanto delle operazioni molto limitate e mirate, che non configurano

risposta del Ministro, soprattutto del tono che ha usato e dell'approccio razionale ad un problema che ha - come tutte le crisi internazionali - innumerevoli aspetti da da tenere sotto controllo: l'unità del Paese, la stabilizzazione del Governo libico e, contemporaneamente, l'impegno sul piano umanitario, che si potrà poi

dovrebbe agire in modo unitario e noi stiamo provando a farlo. Purtroppo, qualche anno fa l'azione europea non è stata un'azione lungimirante verso la Libia e sono convinto che adesso lavoreremo con maggiore sono parzialmente insoddisfatto della risposta del Ministro, nel senso che alcune risposte non sono state date. Siamo di fronte a due scenari: uno è quello siriano, di cui parleremo tra poco, dove c'è un intervento molto efficace, devo dire, da parte della Russia per il ristabilimento di un minimo di equilibrio delle forze in campo. Si potrà dire di tutto del regime di Assad, ma è certo che con l'intervento della Russia c'è stata una compressione del territorio controllato da Daesh. In Libia sembra di assistere ad un ragionevole immobilismo delle cancellerie occidentali

timore che possiamo avere come italiani è che, pur venendoci riconosciuta dalla comunità internazionale la guida di qualsivoglia missione, nelle forme che verranno stabilite, ci sia il rischio che si ripeta l'episodio di Sabrata. Mi auguro che questo non accada. Dalle parole del Ministro non dovrebbe accadere, ma non ne abbiamo le certezza.

lo scenario entro il quale si sta consumando la crisi libica e la relativa posizione italiana. Come si diceva, la posizione francese, nella sua mancanza di ufficialità, rappresenta un rischio, non solo per la mancata attuazione dell'obiettivo condiviso al livello transnazionale del riconoscimento del Governo di unità nazionale, ma anche per l'inconsistenza di una posizione unitaria della Comunità europea, che indebolisce il progetto di stabilizzazione della Libia, la cui priorità è stata ribadita anche a margine del recente Consiglio UE per gli affari interni. voglio innanzi tutto ringraziare il Ministro per il tono, la cautela e il buon senso di quanto gli ho sentito dire, però devo dichiararmi insoddisfatto, perché non ha risposto al quesito se Haftar sia da considerare un nostro alleato o un avversario, non ha risposto al quesito se una missione statica (difendere i pozzi o Tripoli) non sia addirittura più pericolosa che inseguire Daesh, e non ha risposto alla richiesta di un dibattito parlamentare serio e approfondito come quello che c'è stato in Gran Bretagna.

e per il quadro che ha voluto disegnare, certamente non facile e non sereno, di una situazione come quella libica. Ritengo che il percorso che l'Italia sta seguendo sia quello del buon senso e della ragionevolezza

sul Parlamento di Tobruk, affinché, attraverso la sua deliberazione, possa finalmente dare più forza, più slancio e più capacità di azione al Governo che si è insediato. [MAURO

È vero che ogni Paese, pur condividendo gli intenti generali dell'azione che la comunità internazionale si è prefissa in Libia, si muove sulla base dei propri interessi. Sarebbe però importante capire se quelli che sono gli alleati della leva europea e degli accordi internazionali da noi siglati, come gli Stati Uniti,

abbiamo mandato via i dittatori, ma abbiamo creato la destabilizzazione di tutta l'area mediterranea. Ricordo che la Libia, nel periodo di Gheddafi, aveva un reddito *pro capite* di 14.000 dollari,

utilizzare sarebbe quella di dichiararci parzialmente soddisfatti. Dico «parzialmente» perché il Ministro, con grande equilibrio e accortezza, non ha taciuto alcuna delle preoccupazioni di una situazione molto difficile e molto incerta.

Governo in esilio, evocando la formula di una storia europea lontana. È un Governo in cerca del voto di fiducia, ma è un Governo vero e proprio

Sulla base di questa priorità il Governo italiano cerca di reagire a quel clima - come ha detto giustamente il collega Romani - da un lato, di immobilistica stagnazione stagnazione politico-diplomatica e, dall'altro, di ipervivace agilità affaristica. L'Italia non è complice né della prima, né della seconda e mi pare che il Ministro presidi questa linea con adeguata fermezza.

Signor Ministro, vorremmo conoscere le priorità del Governo italiano sulla questione siriana.

che - secondo chi parla - è una pura questione di diritto interno dei siriani, o sconfiggere e combattere il terrorismo internazionale che tocca innanzitutto tutti i Paesi occidentali, noi compresi? Poiché la prima forza che si è schierata e ha fermato l'ISIS sulla linea di Kobane sono stati proprio i curdi siriani, lei è d'accordo ad ammettere una rappresentanza curda al processo negoziale di pace che si svolgerà per la Siria? [ROMANI

la possibilità, per il nostro Paese, di favorire i famosi caschi blu della cultura. Immagino che fossero di presidio, stabilizzazione e anche per lo sminamento, visto che l'Italia ha una straordinaria capacità a questo riguardo. Abbiamo assistito, però, dopo la rioccupazione di Palmira da parte dell'esercito regolare siriano,

alla seconda domanda. Nell'attesa del ripristino dei negoziati di pace a Ginevra, ancora non è chiaro l'atteggiamento finale del Governo italiano. Abbiamo assistito, purtroppo, negli anni passati all'appoggio da parte degli Stati Uniti di alcuni gruppi che si contrapponevano al Governo siriano, ma in Siria non c'è solo Daesh, che occupa una buona parte del territorio, ma c'è soprattutto al-Nusra, la costola siriana di al-Qaeda. Non saprei chi scegliere tra i due gruppi terroristici. Tutte le armi, anche molto raffinate, anticarro e antiaerei, fornite dagli americani ad alcuni gruppi che si contrapponevano al Governo di Assad, sono finite nelle mani di al-Nusra. Abbiamo, quindi, indirettamente alimentato gruppi terroristici.

incredibile, ma divisa in due parti con centinaia di migliaia di cittadini che soffrono per questa divisione. Siccome sembra essere in atto un'offensiva del Governo siriano per la possibilità di rioccupare

*(PD)*. Signor Ministro, la questione drammatica della guerra civile e della crisi siriana insiste in un quadrante decisivo dello scacchiere internazionale che ha enormi implicazioni geopolitiche a livello mondiale. E questa crisi è un fattore che riacutizza i nervi scoperti delle relazioni internazionali tra le potenze regionali e internazionali. La crisi geopolitica porta con sé la necessità di ristabilire una nuova stabilità nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente e poi soprattutto due grandi questioni, la cui soluzione ha a che fare con la tenuta stessa dell'Europa e del suo percorso di integrazione. Una è quella dei flussi migratori legati alle guerre. Le cifre parlano di 7 milioni di sfollati, di cui 4 milioni di rifugiati, la maggior parte in Giordania, in Libano e in Turchia, ma molti - come sappiamo - anche in Unione europea. Vi è, poi, la questione del terrorismo jihadista, l'ingresso di Daesh nel territorio siriano. Per fortuna, notizie delle ultime settimane sono le vittorie che l'hanno risospinto verso l'esterno, ma anche il posizionamento di al-Qaeda. Dal marzo 2011 vi è una rivolta contro il regime di Bashar al-Assad, che si è macchiato di persecuzioni molto gravi contro la popolazione (250.000 vittime),

colloqui di pace, coordinati dall'inviato ONU Staffan de Mistura, che hanno messo al centro un documento con

nuove elezioni libere. A margine, c'è anche una questione molto importante, quella curda, la cui risoluzione è fondamentale per gli esiti positivi

Signor Ministro, uno dei nodi più delicati dell'*impasse* siriana resta quello del flusso costante ed emergenziale dei migranti. È questo uno degli argomenti di maggiore attenzione mediatica soprattutto in Europa, anche in ragione dei problemi che sta comportando sul fronte dei rapporti e delle decisioni tra i diversi Stati membri. Sul fronte territoriale, le informazioni sono ancora più confuse, così come il ruolo della comunità europea. Appare, però, chiaro il ruolo determinante della Russia, che, con il suo dispiegamento di forze e il suo supporto strategico, ha sostenuto e rafforzato Assad nel contenimento dell'avanzata non solo delle forze dell'ISIS, ma anche dei gruppi di opposizione nel loro complesso. Ovviamente questo scenario esorcizza di fatto l'ipotesi di una sorta *exit strategy* per Assad, seppur ventilata nelle scorse settimane da alcune indiscrezioni della stampa panaraba. Se sul fronte strategico, però, sembra chiara la posizione russa, di contro vi sono molte difficoltà nell'inquadrare quella della comunità internazionale, anche in ragione delle posizioni talvolta discordanti dei diversi *partner*. Nel frattempo, la situazione nelle aree di crisi continua a essere drammatica drammatica e la popolazione continua a essere stretta nella fame. Una città come Aleppo da mesi è teatro di intensi scontri, nonostante il cessate il fuoco in vigore. In uno scenario complesso come quello attuale, vorremmo tentare di comprendere come stanno realmente le cose e che ruolo ufficiale sta assumendo e intende assumere l'Italia nella comunità europea. innanzitutto vorrei esprimere apprezzamento per il ruolo che l'alto commissario Mogherini ha avuto nella regione, in particolare nel negoziato con l'Iran, che è parte importante del tentativo di stabilizzare la regione, e apprezzamento anche per la prudenza con cui lei, ministro Gentiloni, ha affrontato la questione russa. Ma venendo allo scenario, non mi pare che sia più in discussione la questione di Assad. Se la Siria rimarrà unita, Assad non sarà più il *rais* della Siria. la questione è un'altra. Signor Ministro, non ha l'impressione che il nostro alleato, l'Arabia Saudita, stia rallentando in tutti i modi la resa dei conti delle milizie curde, degli iraniani e dell'esercito iracheno con Daesh, nell'attesa di costruire un forte partito wahabita La seconda questione riguarda un altro alleato. La Turchia combatte i combattenti curdi, che sono i più attivi contro Daesh. Inoltre, gli accordi che sono stati presi con l'Unione europea parlano di zone proprio alla frontiera per accogliere i rifugiati. Mi sembra, con ogni evidenza, un tentativo di combattere ulteriormente i curdi, di mandare lì l'esercito turco e di riguadagnare quel terreno alla Turchia, che era alleata con forze che non erano molto lontane da Daesh e che trafficava con Daesh, per farle rimettere un piede in quella zona delicata, ai danni dei curdi. Vorrei sapere cosa ne pensa.

fonti del regime di Damasco danno però annunci di un'ulteriore e necessaria fase di colloqui con i movimenti di opposizione, proprio in virtù delle proposte di cambiamento di carattere costituzionale della bozza di piano di pace presentata a Ginevra. Da fonti ONU pare ci siano stati la conferma di questo accordo raggiunto dalle parti per una transizione al fine di definire una nuova forma di Governo e, quindi, la sollecitazione

che sembrano intenzionati a incrementare la propria presenza in Siria al fine di rafforzare la lotta ai militanti dell'ISIS, e alla Russia, che sembra stia preparando una nuova risoluzione da presentare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di fronte a questo ipotetico scenario, vorrei conoscere il ruolo dell'Italia e la nostra azione.

Il 24 marzo scorso l'esercito siriano e i suoi alleati hanno finalmente cacciato l'ISIS da Palmira, avviando il processo di sminamento dell'area e il recupero dei monumenti. Rimane però il nodo politico della guerra in Siria, che non è stato ancora sciolto. I negoziati di pace iniziati a Ginevra hanno escluso una delle forze più importanti, cioè quella dei curdi, i quali - come spiegato in occasione di un incontro in Commissione affari esteri con il Presidente del Parlamento della Regione del Kurdistan sono gli unici non solo a lottare contro il Daesh, ma anche ad aver elaborato una chiara posizione per la definitiva soluzione del conflitto, proponendo un modello di cantonalismo originale ed efficace nell'attuale sistema mantenendo rapporti sia con il Governo siriano che con le fazioni ribelli. La loro esclusione ci dà l'impressione di lasciare troppa mano libera alle pretese della Turchia. Forse sarebbe giunto il momento di cambiare strategia, immaginando un coinvolgimento internazionalistico e sovranazionale riguardo al conflitto siriano, dopo anni di illegale sostegno alle milizie armate dei ribelli che hanno generato solo *caos* e distruzione. Con riferimento al negoziato di pace, chiedo di conoscere la posizione del nostro Governo circa la decisione di escludere i curdi dal tavolo del negoziato, nonostante sinora siano stati coloro ad aver combattuto contro l'ISIS, difendendo Kobane a caro prezzo. Ricordo che la questione siriana è la causa principale dell'ondata migratoria che sta mettendo in crisi le politiche europee, come dimostra la posizione austriaca sul valico del Brennero. non ritiene, quindi, che la mancanza di dialogo con il Governo siriano renderà sempre più difficile la gestione sia del flusso dei migranti che della sicurezza dei nostri territori? Visto che è all'ordine del giorno il ritrovamento di documenti siriani falsi, senza la collaborazione siriana sarà difficile contrastare questo fenomeno. Chiedo, quindi, se il Governo abbia valutato la possibilità di ripristinare le relazioni diplomatiche con la Repubblica araba siriana, nonché l'ipotesi di aprire l'ambasciata Grazie, signor Presidente. Ginevra ristagnino, e questa è la sensazione che si è avuta anche ieri. Del resto, la tregua fatta a fine febbraio era, appunto, una tregua e non un inizio di pace,

la città di Aleppo, che è divisa in due. D'altra parte, è stata evocata da molti la questione dell'anticurdismo pregiudiziale della Turchia, che ha reso tutto più difficile. D'altra parte, per note ragioni, evocate anche queste dai colleghi, i Paesi europei sono sotto il peso della pressione demografica e dell'esigenza di doverla in qualche modo trattenere attraverso accordi con la Turchia. Allora, da questo punto di vista, è il momento di scegliere fra le priorità della nostra diplomazia. della nostra diplomazia. C'è una posizione americana e occidentale, per la quale Assad non è più proponibile come Governo; c'è, anche se gli viene attribuito dai commentatori - non sempre Putin in prima persona lo precisa - un "assadismo" pregiudiziale da parte di di Putin, che è sceso in campo alla fine dell'anno scorso e che - non c'è dubbio - sarà uno dei protagonisti della trattativa di pace, se riuscirà a Al momento, lo stallo di Ginevra è da registrare con molta preoccupazione, e forse era stata troppo enfatizzata come pace la tregua di fine febbraio.

credo che negli ultimi sette o otto mesi l'approccio di buona parte della comunità internazionale alla crisi siriana sia andato chiarendosi

Cosa abbiamo sostenuto negli ultimi due o tre anni? Abbiamo sostenuto che certamente bisognava accompagnare la transizione in Siria, perché non possiamo dimenticare le responsabilità di Bashar al-Assad in quella che è stata la catastrofe umanitaria più grave degli ultimi vent'anni. Parliamo di centinaia di migliaia di morti. Parliamo di quello che ha provocato lo sfollamento di milioni di persone, l'origine principale dei flussi migratori nella rotta balcanica. Queste sono responsabilità che il dittatore siriano porterà con sé. era una posizione che, pur non ignorando tutto questo, metteva in guardia dall'illusione che, con una spallata militare, si sarebbe potuta risolvere la crisi siriana e anzi avvisava che, solo con questa impostazione, c'era il rischio che, travolgendo quel regime, si ricreasse un vuoto e che esso venisse di nuovo riempito, com'era accaduto dodici anni prima in Iraq, da qualcosa che assomigliasse molto da vicino a Daesh e alla crescita del terrorismo. Ora, direi che su questa linea - molti la sintetizzano con l'espressione «*Assad change, not regime change»*, ma lasciamo stare le formule diplomatiche - c'è una larga convergenza della comunità internazionale. Credo che di nuovo siamo stati abbastanza pionieri nel dire che certamente il ruolo della Russia conteneva dei pericoli, in termini di ingaggio diretto tra superpotenze e di un atteggiamento di sostegno fino alla morte alla posizione di Assad, ma esso poteva anche essere un'occasione costruttiva. Alla fine, almeno negli ultimi mesi, si è vista una io non discuto che ci sia stato un ruolo importante della Russia nel sostenere Assad, ma discuto che la Russia abbia un interesse a sostenere questo regime per credo che oggi abbia un interesse a favorire una transizione. E la transizione, senza creare un vuoto, deve naturalmente superare anche la persona del dittatore, cui non può essere affidato probabilmente il futuro della Siria.

di lavoro sulla Siria, spesso con una collaborazione di posizioni e di opinioni. Ma, nonostante questo, non dobbiamo illuderci di essere nel contesto di trent'anni fa, in cui un accordo tra russi e americani metteva la camicia al mondo, delle posizioni di diversi altri Paesi. È stata citata l'Arabia Saudita, ma cose simili, sia pure completamente diverse, si potrebbero dire dell'Iran. Non è che, se la Russia decide una cosa, l'Iran rinuncia ai propri interessi nazionali o viceversa nel caso dell'Arabia Saudita. Quindi, la prima difficoltà è una è una prova di un multilateralismo complicato. Non è di nuovo un gioco di due superpotenze che aggiustano il mondo. Quanto alla seconda difficoltà, la situazione la situazione sul terreno aveva dato vita a un mezzo miracolo, diciamo la verità. A fine febbraio nessuno si illudeva. Ricordo che entrammo in una riunione che durò otto ore in un albergo di Monaco

c'è stata la cessazione delle ostilità da quel 27 febbraio, con una riduzione dei bombardamenti e della violenza attorno al 70-80 per cento; con l'accesso umanitario a centinaia di migliaia di persone sotto assedio e che stavano morendo di fame; con risultati molto importanti; con l'avvio di negoziati cosiddetti di prossimità, nei quali le diverse parti sono istanze diverse, non si siedono attorno a un tavolo e l'inviato delle Nazioni Unite, il nostro Staffan de Mistura, fa la spola tra le diverse parti. Tuttavia, non dobbiamo nasconderci che nelle ultime due o tre settimane questi fatti positivi sviluppati sul terreno sono messi in crisi. Purtroppo il livello di violenza è cominciato ad aumentare deriva da tante ragioni che sarebbe troppo lungo descrivere. Ma il problema di fondo è che, essendosi dichiarata la cessazione delle ostilità (fatte salve le attività contro Daesh e al-Nusra), ed essendo al-Nusra posizionata in territori nei quali la sua presenza è molto intrecciata a quella di forze dell'opposizione siriana, alla fine, combattendo al-Nusra, molto spesso si sono ingaggiati di nuovo combattimenti tra le due parti, governative e di opposizione siriana. E questo ha ridato vita a una spirale di violenza. Bisogna stare molto attenti. Quindi, la decisione che sta maturando è - credo nei prossimi dieci giorni - di riunire di nuovo la conferenza ministeriale del gruppo di sostegno alla Siria per cercare di ridare impulso a un processo. Innanzitutto, il cessate il fuoco per ragioni umanitarie in questo momento è quasi più importante dei negoziati. I negoziati avranno bisogno di tempo per produrre risultati. Se però si chiudono i corridoi umanitari, se il regime torna a un atteggiamento di chiusura verso i convogli umanitari, allora veramente torniamo alla casella di partenza. Credo, quindi, che serva rapidamente un rilancio.

dei curdi siriani, nella dinamica negoziale? L'Italia è favorevole, diversi Paesi sono favorevoli, mentre altri sono - come potete immaginare - radicalmente contrari. L'inviato delle Nazioni Unite ha compiuto molte acrobazie, nel senso che ai ai colloqui di prossimità partecipano, sia pure con una partecipazione definita di secondo livello, anche esponenti dell'opposizione siriana, visto che c'è da parte di alcuni attori fondamentali un'opposizione radicale, che ben conoscete, a una partecipazione a pieno titolo. Se però volete conoscere la nostra posizione, quella italiana, noi riteniamo che certamente abbiano svolto e svolgano un ruolo e certamente vadano coinvolti nel processo negoziale. Quanto al tema dell'UNESCO e di Palmira, il 13 aprile

risanamento, alla ricostruzione e alla riprotezione del sito archeologico, che questa missione sarebbe partita quando le condizioni di sicurezza lo avrebbero consentito. è una valutazione che farà l'UNESCO, e noi ci auguriamo che questo sia possibile in tempi rapidi. Infine, uno degli interroganti ha parlato delle nostre relazioni diplomatiche con la Siria. È chiaro che noi non possiamo non avrebbe senso politico - ristabilire pienamente delle relazioni con un regime di cui predichiamo la necessità di essere superato con una transizione, non di essere travolto da *raid* aerei. l'oggetto del negoziato di Ginevra sono i diciotto mesi di transizione, al termine dei quali tutti pensano che il *leader* della Siria non possa essere Bashar al-Assad,

sia facile che in tale contesto egli pronunci queste parole, ma penso sia un interesse comune in cui addirittura russi e americani potrebbero essere al lavoro insieme per favorire una transizione.

del tutto: abbiamo un incaricato d'affari che mantiene rapporti con la Siria e che opera da Beirut, in Libano, e che quindi può essere comunque utile per questioni umanitarie o che riguardano cittadini italiani. C'è un filo che non si è del tutto spezzato, ma che oggi non è immaginabile ritrasformare in piene relazioni diplomatiche.

le cancellerie occidentali e le forze di opposizione, visto che - come ha giustamente detto il Ministro - sono tutte mischiate e anche ISIS è avvenuto su territori dove non c'erano contrapposizioni tra il Governo regolare di Assad e

c'è stato l'inserimento di 250 militari statunitensi in Siria con proteste del Governo di Damasco, non si capisce se si voglia continuare in quella politica di aiuto e anche di fornitura a gruppi di opposizione e come ciò possa essere compatibile con l'effettiva guerra al terrorismo, che è fatto non solamente dal gruppo di Daesh, ma anche da al-Nusra. Mi sembra, quindi, uno scenario particolarmente complesso, dove forse anche per il Governo italiano è più complicato dare risposte più precise.

ribadendo quello che penso sia un punto fondamentale della nostra dottrina politica, che vale per la Siria ma per tutta l'azione nei confronti del Mediterraneo, ovvero che non ci possono essere soluzioni militari senza

centro la transizione democratica in Siria al termine dei diciotto mesi. Penso, infatti, sia obiettivo nostro andare oltre la tenaglia tra dittatura e fanatismo, fare in modo che la nostra politica estera sia improntata a un realismo che, però, abbia al centro l'impegno per la sicurezza e la stabilità, ma anche, come monito fondamentale, per la transizione democratica delle regioni mediorientali e mediterranee. [DI Signor Ministro, la ringrazio per quanto ha voluto condividere con noi, rimarcando ancora una volta l'attenzione che lei riserva alla tematica, soprattutto sul versante umanitario. Sappiamo che la Siria sembra essere diventata la proiezione in scala degli attuali rapporti di forza geopolitici e il ruolo della Russia ne è forse l'espressione più chiara. È per questa ragione che una certa confusione di approcci dell'Unione europea rappresenta purtroppo un pesante limite, soprattutto perché continua solo a essere accostata alle sanzioni contro il Governo siriano, che, stando proprio alle posizioni dei detrattori, hanno il merito solamente di incrementare il flusso dei migranti verso l'Europa. Siamo certi che quanto da lei evidenziato possa essere uno spunto di riflessione interessante per le determinazioni future. sono soddisfatto per la ricostruzione dello scenario che lei ha fatto e per il chiarimento sull'apertura dell'Italia all'inserimento dei curdi nel negoziato. Trovo che non abbia risposto sulla questione più spinosa, e cioè sull'atteggiamento di due alleati dell'Italia, la Turchia e soprattutto l'Arabia Saudita, che - secondo molti osservatori - stanno portando per le lunghe la vicenda e stanno sostanzialmente dando ossigeno e tempo a Daesh.

lo stato delle trattative in seno ai colloqui di pace. In modo particolare confidiamo - è quello che poi oggi è stato evidenziato anche a livello di Nazioni Unite - nell'insistenza a voler subito riattivare il comitato internazionale di sostegno alla Siria da parte italiana per potere proseguire sulla strada che, con tutte le difficoltà esposte, penso sia oggi l'unica percorribile per cercare di dare sicurezza a una situazione che guardi innanzitutto agli aspetti umanitari, ma anche in

Da quello che ho potuto capire, l'Italia ha assunto una posizione molto mite e tiepida nei confronti dei curdi. Mi sarebbe, anzi, piaciuto che lei avesse dichiarato chi ha votato contro la partecipazione dei curdi al tavolo di pace, oltre alla Turchia che si deduce abbastanza facilmente.

mi pare più che comprensibile, oltre che apprezzabile, il fatto che il Ministro, ribadendo le responsabilità sotto tanti profili del dittatore siriano, abbia voluto rivendicare una continuità di posizione

Da questo punto di vista, l'Italia non può che rimettersi al tavolo dei due ministri, Lavrov e Kerry, perché ovviamente è da lì che deve il cartellino rosso per Assad. Non è materia di Staffan de Mistura, ma Kerry e Lavrov potrebbero trovare la strada